Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri sera, ha anzitutto stabilito che le dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge concernente il testamento biologico avranno luogo, con trasmissione diretta televisiva, oggi pomeriggio, con inizio alle ore 17. Entro tale orario dovranno pertanto concludersi le votazioni degli emendamenti e degli articoli. La Conferenza dei Capigruppo ha poi approvato il calendario dei lavori dell'Assemblea per le prossime due settimane. Nella seduta pomeridiana di martedì 31 marzo sarà posto all'ordine del giorno il disegno di legge recante disposizioni in materia di usura. A partire dalla seduta antimeridiana di mercoledì 1° aprile sarà esaminato il decreto-legge in materia di produzione lattiera, già approvato dal Senato, ove modificato dalla Camera dei deputati. Nel corso della prossima settimana saranno inoltre discusse ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione e, nella seduta antimeridiana di giovedì 2 aprile, mozioni sul clima. Nelle sedute della settimana successiva, dal 7 al 9 aprile, sarà discusso il decreto-legge sul sostegno ai settori industriali in crisi, in corso di esame presso la Camera dei deputati. Nella seduta antimeridiana di mercoledì 8 aprile, alle ore 12, si procederà alla votazione a scrutinio segreto con il sistema elettronico per l'elezione di due componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Per i decreti-legge previsti dal calendario si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Resta confermato che l'Assemblea non terrà seduta nella settimana successiva alle festività pasquali. Nel corso di tale settimana le Commissioni potranno convocarsi in relazione ai rispettivi programmi dei lavori. Alla ripresa dei lavori dell'Assemblea saranno esaminati il decreto-legge in materia di atti persecutori - attualmente all'esame della Camera dei deputati, in scadenza il 25 aprile nonché il disegno di legge collegato sul federalismo fiscale, secondo il calendario che sarà stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, da convocare prima della sospensione dei lavori. In sede di programmazione sarà inoltre considerato il disegno di legge collegato in materia di internazionalizzazione imprese ed energia.

La seduta è ripresa.

precisamente, nel parere proposto dal relatore il 25 febbraio 2009 si ribadisce che se fosse negato il carattere vincolante di una dichiarazione, che per definizione non può essere confermata da un soggetto che abbia perso la capacità di intendere e di volere,

e, a titolo personale, sono in totale disaccordo per i princìpi generali che sono stati già enunciati poc'anzi. Quando Quando in una norma si confondono i desideri con il piano giuridico, le aspirazioni con una regola, allora significa veramente porre in essere una legge che non ha alcun significato.

è esattamente contrario all'emendamento 4.23, di cui sono primo firmatario. Volevo solo ricordare che la Commissione giustizia, con l'unanimità l'unanimità di tutte le forze politiche, ha sostenuto la necessità di rendere giuridicamente vincolanti le dichiarazioni. Ora sarebbe una sorpresa notevole se in Aula i membri della Commissione giustizia, già così convintamente concordi, dovessero cambiare idea e votare in senso contrario a quello che in coscienza avevano votato all'interno della Commissione. Signor Presidente, credo che i colleghi che sono intervenuti difendendo il testo originario avrebbero ragione se si passasse al testo opposto, che poi è previsto in un successivo emendamento, nel quale si dice che le dichiarazioni non sono obbligatorie né vincolanti. Noi ci fermiamo al «non sono obbligatorie» e rimandiamo all'articolo 9. 9. Questo per chiarezza, perché abbiamo previsto un margine per il medico per poter intervenire a favore del paziente nel caso ci siano delle evenienze, anche di carattere scientifico, che si verifichino dal momento della dichiarazione al momento della scelta, e questo margine lo vogliamo preservare con chiarezza. Quindi ci fermiamo al «non obbligatorie» e non invertiamo un criterio,

perché si fanno fare delle dichiarazioni che non hanno alcun senso, di cui altre persone possono fare quello che vogliono e considerarle carta straccia. Prendiamo atto di questa posizione del Governo e della maggioranza. Noi voteremo a favore dell'emendamento 4.23,

risulterebbe incomprensibile per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.17 (testo 2) che abbiamo votato poco fa. votato poco fa. Infatti, con quell'emendamento avete approvato una norma in base alla quale la dichiarazione anticipata di trattamento produce gli effetti indicati all'articolo 7,

non so se l'Assemblea si sia resa conto davvero di quanto accaduto con la votazione degli emendamenti precedenti. Mi rivolgo soprattutto ai colleghi della maggioranza:

che seppure un individuo ritenga, esercitando la propria libertà, di scrivere, per il momento in cui non sarà più capace di intendere e di volere, e di consegnare nelle forme prescritte le dichiarazioni anticipate di volontà, tali dichiarazioni non conteranno assolutamente nulla.

finzione non regge: non regge in quest'Aula, ma non regge neanche nei confronti del Paese! Avete spiegato agli italiani che state scrivendo norme sul testamento biologico. State spiegando agli italiani che la loro volontà non conta niente. Il contrasto con l'articolo 32 della Costituzione è, a questo punto,

sua essenza e nella sua logica, non è mai cambiato. Quando abbiamo scritto che le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono vincolanti, fatto salvo

neanche cercare di renderle più cogenti e più chiare ed avere una legge che non dia adito ad altri procedimenti giudiziari o ad interpretazioni. Non ha senso quanto è scritto nelle dichiarazioni, perché non sono vincolanti. Sono inutili!

è una precisazione al comma 3 dell'articolo 4 e identifica, anche nello spirito di quello che lei ha detto poc'anzi su un altro tema e su un precedente emendamento, relatore Calabrò, la volontà di meglio qualificare e confinare, nel senso di porre limiti,

il testo del terzo comma dell'articolo 4, ma precisa che «in caso di mancato rinnovo e della successiva perdita della capacità di intendere e di volere, il medico curante assume le proprie decisioni di ordine terapeutico con un'attenta valutazione della volontà espressa dal soggetto».

*(PdL)*. Credo che occorra prendere coscienza che le dichiarazioni anticipate non rappresentano un atto ordinario, o comunque di diffusa applicazione, ma hanno un contenuto straordinario ed impegnativo, al di là delle battute polemiche sollevate prima dall'opposizione,

esistono anche altri modelli. Credo sia ragionevole e del tutto fondata la previsione che queste dichiarazioni debbano avere un minimo di serietà e di solennità. Questo vale per le dichiarazioni che vengono rese in senso positivo o per le modifiche. Voglio anche ricordare ai colleghi che se c'è un effetto

non è così per la revoca, perché non si può impedire né si può pensare che una persona che ha rilasciato le dichiarazioni nelle forme previste di atto, nella stessa forma, per poterle revocare. Immaginiamoci una situazione particolare in cui non ci sia il medico, non ci sia la possibilità di scrivere o non ci sia la possibilità di redigere un atto del genere. Una persona che volesse revocare in quel momento le proprie dichiarazioni non potrebbe farlo. Allora, mi sembra del tutto logico e coerente, anche con il sistema giuridico (ma soprattutto con la coscienza di tutti noi), che per la revoca ci sia libertà di forma. La revoca deve essere espressa, non può essere presunta, ma deve poter deve poter essere resa in forma libera, cioè senza i vincoli previsti da questo articolo.

surreale. Se capisco bene l'emendamento, noi abbiamo appena deciso che le dichiarazioni che vengono rilasciate con questa procedura (addirittura il collega Massidda voleva che si andasse dal notaio) degli orientamenti su cui poi il medico curante deciderà. Nulla mi impedisce di dire la mia opinione al medico curante con una cartolina postale che gli spedisco qualche giorno prima, non capisco cosa cambi ai fini dell'efficacia. Tuttavia, se con una procedura così come viene definita io sono costretto ad andare dal medico di medicina generale e a portare un testimone per decidere chi è il mio fiduciario, e se ora

Signor Presidente, molto brevemente: questo è il discorso più strampalato dal punto di vista giuridico che ho sentito svolgere da una persona esperta di diritto, ossia da un notaio. Senza vincoli di forma significa che la revoca può essere fatta anche oralmente. Non so come un notaio possa ritenere che si possa revocare un atto che ha un suo contenuto formale definito con un atto privo di forma. È il discorso più strampalato che abbia mai sentito pronunziare.

intervengo solo per richiamare l'attenzione del relatore e del Governo sulla portata normativa di questo emendamento, che si colloca dentro l'ormai esplicito tentativo

con qualsiasi forma. Per chi ha un minimo di cognizione sulla forma di un negozio giuridico, ciò significherà che la dichiarazione anticipata di trattamento sarà revocabile anche verbalmente:

molto seria e, poiché non mi presto ad operazioni funzionali alla cosiddetta eterogenesi dei fini, cioè ad affidare ad un magistrato l'interpretazione della volontà postuma del soggetto in ordine ad una dichiarazione di revoca che non ha i requisiti di sostanza e di forma della dichiarazione anticipata di trattamento, questa idiozia non la voto! Presidente, non ci prestiamo al gioco di chi vuol fare credere che l'aver detto che le DAT non sono obbligatorie significa togliere ogni valore a queste dichiarazioni,

spiegata per bene. Chiedo comunque al collega Pastore di ritirare l'emendamento 4.140, come atto di buona volontà nei confronti di argomentazioni che hanno un senso.

che, quando il punto verrà attentamente considerato, si trarranno conclusioni diverse, anche da parte dei colleghi che hanno usato espressioni un

sono però convinto che, una volta meditata la questione, su questo punto magari i colleghi della Camera faranno una riflessione ulteriore. Accolgo quindi l'invito del mio Capogruppo vicario e ritiro l'emendamento 4.140, pur confermando

Presidente, desidero scusarmi con il senatore Pastore, ma il termine «idiozia» non era rivolto a lui, né alla proposta.

abbiamo proposto lo stralcio del comma 6 dell'articolo 4, che vado a leggere anche perché forse può essere collegato all'ultima fase del dibattito che ci ha occupati. Si dice al comma 6 dell'articolo 4: «In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato,» qualsiasi esso sia - «la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica». Ancora una volta, si certifica il fatto che ci viene detto qualcosa con ampio respiro retorico in quest'Aula, ma poi si scrive il contrario,

avere una delucidazione dal relatore. Nel caso in cui un testimone di Geova dovesse trovarsi in condizioni di pericolo immediato e dovesse, per motivi religiosi (discutibilissimi, per carità), carità), aver scritto e portare su di sé la esplicita richiesta di non subire una trasfusione di sangue,

che una legge possa prevedere trattamenti sanitari obbligatori o limitazioni ai diritti fondamentali di libertà della persona, anche se emanata in violazione dei princìpi contenuti nella Costituzione stessa. Si può facilmente prevedere che anche sulle definizioni di trattamento sanitario, terapeutico e sostegno vitale si formerà un contenzioso che finirà con l'essere oggetto di ricorsi al giudice ordinario e alla Corte costituzionale. Per fortuna, in questo contesto, in cui la Costituzione appare svilita da interpretazioni che francamente lasciano sbigottiti i giuristi e devono preoccupare chi ha a cuore la democrazia, esiste la Corte costituzionale. Corte che da pochissimo tempo, a fine dicembre 2008, con la sentenza n. 438, 438, ha ribadito che è imposto l'obbligo per lo Stato di consentire a ciascuno l'espressione delle proprie volontà in merito ad ogni tipo di trattamento sanitario, garantendone la vincolatività, trattandosi di un vero e proprio diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione. Analogamente, la Corte suprema di cassazione, con la sentenza, a Sezioni Unite penali, del 21 gennaio 2009, n. 2437, ha ribadito che il bene della salute è tutelato dall'articolo 32 non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo. Allora, se questi sono i principi a cui occorre uniformarsi per il rispetto dei principi della Costituzione, che la Corte costituzionale e la Corte di cassazione a Sezioni Unite, vale a dire i massimi vertici della giurisdizione, ci propongono e di cui noi parlamentari per primi dobbiamo necessariamente e istituzionalmente fidarci, il commento all'articolo 4 diviene veramente imbarazzante. La norma, oltretutto, per il combinato disposto degli articoli 4 e 7, propone una irragionevole violazione di diritti fondamentali anche sotto un altro profilo, poiché non dà riconoscimento all'irrinunciabile diritto del medico curante all'obiezione di coscienza, attraverso la previsione di obblighi per le strutture sanitarie, di sostituzione del medico obiettore. E come escludere poi che il medico possa ritenere di disattendere la norma così approvata, se in coscienza ritenesse che la volontà del proprio paziente debba essere rispettata essendo ciò previsto dalla Costituzione? Cosa accadrà in tali casi sotto il profilo della delazione, della denunzia e dell'autodenunzia penale? Quali e quanti conflitti umani, giudiziari, laceranti? Quindi il comportamento del medico rispetto l'attuazione delle direttive anticipate creerà drammi, con nuove rappresentazioni pubbliche, e ricorsi che trasferiranno al giudice la decisione finale sulle volontà di fine vita, esattamente quello su

che la legge, così approvata, sarà inutile, dannosa e semplicemente disumana.

Tale articolo interviene sulla forma, le modalità e la durata delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Per la verità, l'articolo era entrato in Commissione in forma diversa dalla formulazione che è venuta all'attenzione dell'Aula e che stiamo discutendo e probabilmente, fra tutti gli articoli di questo disegno di legge,

la mancata conferma del vincolo delle dichiarazioni non vuol dire assolutamente che le dichiarazioni anticipate non verranno rispettate, che la volontà del soggetto non viene rispettata. Anzi, è una maggiore tutela e una maggiore prerogativa per la sua vita. Provocatoriamente vorrei ricordare a chi ha sollevato questa polemica che ci sono Paesi, per esempio gli Stati Uniti, dove la gente si fa ibernare nell'attesa e nella speranza che i progressi della scienza possano un giorno permettere di intervenire sul loro cadavere. La durata, che era stata prevista in tre anni, è stata portata a cinque. Ero d'accordo con il senatore Pastore nel rendere le modalità di revoca delle dichiarazioni anche più snelle, più semplici, ma concordo con l'intesa che è stata trovata nel Gruppo di ritirare quell'emendamento. L'informazione che viene data al paziente dal medico di fiducia deve essere puntuale e completa prima della sottoscrizione delle dichiarazioni.

Viene stabilito, infine, che le DAT devono essere inserite nella cartella clinica e che chiaramente, come riconfermato anche poco fa dal senatore Rizzi, non hanno valore nei casi di urgenza oppure quando il soggetto versa in un imminente pericolo di vita. Quindi, signor Presidente, dal momento che l'articolo 4 è perfettamente in linea e in armonia

Presidente, onorevoli colleghi, sfigurato dalla modificazione dell'articolo 4, il provvedimento in esame stabilisce in modo pressoché definitivo che una legge sul testamento biologico si configurerà come una legge che impedisce il testamento biologico. Per contrastare con l'azione del protagonismo civile questo fenomeno di proibizionismo, gruppi di cittadini, liberi e indipendenti, hanno cominciato in tutta Italia a raccogliere le dichiarazioni anticipate di trattamento. È già avvenuto in molte città; ieri a piazza Navona, alla corsia Agonale, quindi davanti al Senato, in meno di due ore, mentre il Senato disponeva della legge,

ma ripone fiducia nell'azione della libera cittadinanza che non rinuncerà nel prossimo futuro, fino a che il provvedimento non avrà il suo compimento alla Camera, a raccogliere le firme sulle dichiarazioni anticipate di trattamento per dimostrare che, se il Parlamento è sempre più orientato a scrivere una legge proibizionista, la cittadinanza, secondo il proprio libero intendimento, testimonia una decisione nettamente contraria.

Ricordo ai colleghi che i tempi dei Gruppi di opposizione si sono esauriti; quindi, pregherei loro di essere estremamente concisi

Presidente, un parere della 1a Commissione ci invita a riformulare con maggiore correttezza una parte dell'emendamento 5.100. Quindi vorrei rileggerlo in maniera tale da essere più chiaro: "Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adotta le linee guida nell'ambito delle quali le Regioni provvedono affinché sia assicurata l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente". dal senatore Astore

Il Parlamento, per la prima volta, può dichiarare che questo è un LEA, al di là delle competenze socio-sanitarie o degli ammennicoli vari che la legislazione corrente sta portando avanti con alcune

anche la nuova identità familiare e concetti di abbandono che si stanno verificando nel nostro Paese. Io conosco famiglie, mogli e mamme disperate. È gente che non ha i soldi per poter curare

l'Associazione Luca Coscioni e i Radicali italiani faranno una manifestazione a favore dell'eutanasia e del testamento biologico, più che mai oggi importante dopo il voto espresso da questa Aula. Essi consegneranno le firme al Parlamento

«Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta le Linee Guida nell'ambito delle quali le Regioni provvedono affinché sia assicurata l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente». del Governo è conforme a quello del relatore, ma la rilevanza del tema sollevato poco fa dal mi porta ad una breve considerazione. L'assistenza domiciliare è invero un dovere del nostro Servizio sanitario nazionale.

domiciliare e quindi a sostegno del decisivo ruolo delle famiglie con riferimento alle persone che si trovano in questa condizione.

che ovviamente non consente la diffusione della medicina nel territorio e la diffusione di quelle prestazioni che lei ha giustamente invocato a proposito delle famiglie che sostengono amorevolmente una persona in uno stato vegetativo persistente.

riconvertire, riqualificare, talvolta anche soltanto chiudere strutture che consentano di liberare risorse per i servizi socio-sanitari assistenziali nel territorio. Non è un caso che poi, se si confronta soprattutto la forma plurale di sostegno alla non autosufficienza nelle aree efficienti del Centro-Nord, nell'Emilia-Romagna, nella Toscana, nel Veneto, nella Lombardia e nel Piemonte con le condizioni di inefficienza del Centro-Sud si una differenza spaventosa. I livelli di servizio domiciliare sono proprio la misura della diversa efficienza dei due modelli. È per questo che le rispondo che il tema non è affidato ad una norma manifesto,

il problema non è di soldi, ma di qualità nella gestione del servizio sociosanitario e di coraggio degli amministratori regionali nel rapportarsi con le loro comunità e nello spiegare che la chiusura di quell'ospedale marginale

questo nuovo articolo non prevede l'introduzione dell'assistenza ai soggetti in stato vegetativo tra i livelli essenziali di assistenza.

Guida le Regioni dovranno provvedere ad assicurare l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente. Quindi, è una norma che non dà una risposta immediata e che, come sempre succede, non si sa quando entrerà in vigore.

Grazie,

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

5a Commissione ha fatto il suo lavoro e ha detto che questo articolo non era coperto finanziariamente. Quale è stata invece la risposta della maggioranza su un articolo che poteva essere completamente condiviso?

che l'indicazione di cosa sta e cosa non sta dentro i livelli essenziali di assistenza è contenuta in un decreto legislativo che ancora deve essere emanato.

per una ragione: all'interno delle risorse assegnate alla Regione Veneto sulla base di modelli organizzativi, nell'ambito di ogni unità sanitaria locale la maggior parte della spesa è dedicata ai servizi territoriali, quindi meno del 50 per è dedicato a strutture ospedaliere. Ciò è accaduto perché evidentemente in quel caso si è compiuta la scelta di concentrare la risposta ai malati acuti in strutture in cui, concentrandosi a loro volta le professionalità e le tecnologie in base a questa scelta, è stato possibile organizzare per tutte le forme di non autosufficienza un'offerta plurale fatta di soluzioni residenziali, semiresidenziali, domiciliari con un grande ruolo del volontariato. tanto più vero quando ci si trova di fronte ad una situazione di stato vegetativo persistente, ove quasi sistematicamente il ruolo delle famiglie è assolutamente determinante talmente generoso, vorrei dire eroico senza retorica, che deve essere primariamente sostenuto e supportato. Ed è così. Qual è il problema in una Regione? Mi faccia riproporre l'esempio facile; potrei farne altri, ma quello della Calabria è disgraziatamente troppo facile. BRUNO *(PD)*.

non c'è nella misura in cui servirebbe, mi consenta, perché la struttura complessiva della spesa socio-sanitaria di quel territorio fa sì che non si possa definire,

e dedicato all'assistenza domiciliare, oltre che a quella - come ho ricordato - nelle speciali unità di accoglienza permanente (SUAP) all'interno delle strutture sanitarie proprio per malati in stato vegetativo persistente. La scelta compiuta è che, nell'ambito delle risorse date, ogni Regione è tenuta a garantire i livelli essenziali di assistenza. Lei non potrà mai inseguire le Regioni inefficienti che, nonostante le risorse teoricamente sufficienti, non compiono il loro dovere di garantire i livelli essenziali di assistenza con altre risorse. Negherebbe proprio l'idea di quel federalismo fiscale che già oggi dovrebbe essere vigente per quanto riguarda la gestione del Fondo sanitario nazionale. *(Applausi dal Gruppo disponibilità di risorse aggiuntive che possa sostituire la mancanza di responsabilità di Regioni inefficienti.

la parola quando ciò non è previsto, naturalmente su quello che ha detto il Governo, Ma se lei mi deve convincere del fatto che le dichiarazioni del Governo riaprono un dibattito a tempi esauriti, le dico che non è così secondo la Presidenza. Le concedo tuttavia la parola secondo la mia procedura di disciplina del Regolamento, che è cosa diversa. Mi riferivo semplicemente al fatto che stiamo continuando a svolgere una discussione che prevede, anche a tempi esauriti, qualche brevissima dichiarazione.

testo originario apprezzato da tutti i Gruppi di opposizione e di maggioranza, che diceva che queste prestazioni e questo tipo di attività e di assistenza rientrano nei livelli essenziali di assistenza. La Commissione bilancio - a mio giudizio del tutto correttamente

A partire da questa valutazione della Commissione bilancio, non smentita da nessuno e non smentibile quindi nemmeno dal Ministro, com'è ovvio, perché risulta dagli atti della nostra discussione, non si è provveduto ad apportare al testo la necessaria copertura (probabilmente sarebbe stata possibile una copertura anche molto limitata), ma si è provveduto a smontare il testo, eliminando il riferimento ai livelli essenziali di assistenza. Il senatore Lusi ha semplicemente precisato che

aveva ritenuto la versione originaria di questo testo bisognosa di una copertura finanziaria corretta. Per questa ragione ribadiamo il nostro giudizio negativo. Era molto meglio il testo originario, ma il Governo non ha fatto quello che doveva, cioè appostare una corretta copertura. *(Applausi

all'interno delle abitazioni, negli ospedali o in altre strutture. E se questa figura di fiduciario così impegnato, quindi obbligato a riferire se vengono commessi reati, non riferisce, può incorrere in omissione d'atti d'ufficio? Sarà sanzionato a norma del codice penale? Questa è una figura nuova, che vi siete inventati, e che non c'entra niente con il testamento biologico, ma che dà il senso del modo di procedere: lavorate a caso.

Siete così perseguitati dalla possibilità che si possa legalizzare l'eutanasia in Italia che infilate riferimenti senza senso in ogni parte del disegno di legge.

obiettare al nulla è francamente difficile. Quindi, ritiro l'emendamento.

Presidente, la tentazione che abbiamo in questo momento sarebbe quella di piantare qua tutto e di andarcene di legge è stato svuotato completamente nel dibattito parlamentare. Non solo, e mi rivolgo ai colleghi della Commissione sanità, con cui abbiamo lavorato per parecchio tempo: tutto quel lavoro è stato preso e buttato esattamente nel cestino nel corso dell'esame La maggioranza si è ridotta in un vicolo cieco, in un recinto fondamentalista che veramente non ha alcun senso, quando invece il carattere della moderazione doveva essere quello che guidava la stesura di questa legge per tutti gli italiani. Questo criterio è stato completamente rimandato al mittente e capisco anche perché nell'articolo 6, a questo punto, non si è voluta l'obbligatorietà del fiduciario, che doveva garantire l'alleanza terapeutica. Infatti, se non c'è il fiduciario, l'alleanza terapeutica non esiste, manca uno dei pilastri dell'alleanza terapeutica. Voi non l'avete voluto, ma si è capito perché, di fatto, avete distrutto anche il discorso dell'alleanza terapeutica: non c'è proprio più nulla che regge in questa legge, quindi chiaramente che il fiduciario ci sia o meno non cambia assolutamente nulla. Ciò non toglie la nostra fortissima contrarietà alla rinuncia al fiduciario, per cui voteremo contro l'articolo

Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che sia un po' ingeneroso portare l'argomento a questo Credo invece che, anche in questo caso, si siano recepiti, nella figura del fiduciario, tanti consigli e tanti pareri di tanti colleghi, compresi quelli dell'opposizione. La figura del fiduciario è fondamentale nella legge. esame non è assolutamente svuotato di contenuti, come viene detto, e la vostra stessa battaglia dimostra il fatto che è una legge valida, una legge che dà delle risposte, una legge necessaria nella nostra Nazione. La figura del fiduciario è fondamentale a tutela del cittadino. Il fiduciario ha impegni ben precisi che in questi commi sono ben identificati, per cui rinunciare a tale figura e sminuirla soltanto per una battaglia di contrapposizione politica credo non arrechi alcun giovamento non solo ai cittadini ma nemmeno alla forza politica alla quale lei appartiene,

ha determinato progressivamente, con le modificazioni approvate in Aula, un accrescimento del ruolo del medico e una diminuzione delle volontà del paziente. Il rapporto tra medico e paziente, questa retorica dell'alleanza terapeutica - una vera retorica perché ingannevole - nasconde la sopravvalutazione volontaria del ruolo del medico, il quale diventa arbitro dell'intero quadro della situazione. Il paziente non potrà difendersi perché sarà in condizioni di non poter parlare nel momento in cui si troverà in quelle condizioni, il medico diventa l'arbitro indiscusso della scena. Si è visto che anche il ruolo del fiduciario è svilito e ridotto a poco; quindi, a questo punto, proponiamo, proprio a dimostrazione dello svuotamento del senso del provvedimento, la soppressione dell'articolo 7 per sottolineare,

le parole di un grande uomo. In un'assemblea sull'Unione europea tenutasi in Svizzera davanti a un pubblico variegato e molto agitato, un pubblico

dove l'uomo pensa di essere padrone della donna e dove lo Stato pensa di essere padrone dei suoi cittadini». Ritengo questa frase la più bella definizione d'Europa mai sentita. L'uomo che l'ha pronunciata, Renzo Imbeni, era Vice Presidente in carica del Parlamento europeo. Oggi, con questa legge, caro signor Presidente e cari colleghi, colleghi, stiamo portando l'Italia fuori da questa bella definizione e da questo sogno di Europa dell'amico Imbeni.

quella scienza e coscienza che avete negato ai cittadini e che attribuite solamente al medico o al fiduciario. che a decidere non sono i cittadini, decidete poi che, in caso di conflitto tra fiduciario e medico, decide una commissione di cinque esperti

Dal punto di partenza, volto a negare il diritto ai cittadini, si è arrivati a dare responsabilità indebite ad una serie di categorie

nel momento in cui quest'Aula ha deciso che il principio del *noli me tangere* non esiste più in questo Paese e decide del pari che se sono cosciente posso disporre di me,

mi consentirete nella solennità di quest'Aula, così sorda a qualunque possibilità di suggerimento persino in senso migliorativo rispetto ai pasticci che scrivete, di lasciare agli atti il mio testamento biologico. Lo lascio con grande sofferenza. Lo lascio perché mi sembra l'unico luogo rimasto in cui poter forse consegnare questo documento, che dovrebbe essere un documento così intimo e così privato. Lo lascio perché penso che nel Paese si stia organizzando una vera e propria campagna di disobbedienza civile, lo lascio perché questa campagna rispecchia la dignità che ognuno di noi vuole non solo per sé ma anche per voi, quando ne avrete bisogno.

Voi non ascoltate, non sentite più nulla, come se davvero un dato ideologico, reazionario, avesse offuscato qualunque capacità di dialogo in

Non si tratta di un pericolo remoto. Solo con la sentenza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione del 2009 ha prevalso la tesi secondo cui la condotta del medico, in quanto orientata al beneficio per la salute e non a cagionare una malattia, non può mai dar luogo ad un reato di lesioni volontarie. Ma la medesima sentenza ha una riserva; avverte che l'orientamento giurisprudenziale potrebbe invertirsi proprio a seguito della approvazione della legge sul consenso informato e sulle Così tutte le inevitabili incertezze della legge sul consenso informato si trasformerebbero in pericolosi interrogativi giudiziari penali e si potrebbe procedere per incriminazione per lesioni dolose, quando il pubblico ministero si persuada che il medico ha scavalcato i limiti del consenso informato o, un domani, abbia violato l'articolo 3 delle DAT per non averle considerate con sufficiente attenzione, per non aver spiegato adeguatamente in cartella clinica il perché delle sue scelte, per non aver ben valutato lo sviluppo della scienza medica, o qualora il magistrato ritenga che ci sia stato un assenso di cui all'articolo 2, ma l'informazione preventiva non era adeguata. Per tutto questo, ci sembrava opportuno che le violazioni delle disposizioni formali contenute nella legge siano colpite solo da sanzioni adeguate, ma che resti fermo quanto deciso dalla Cassazione, cioè che il medico agisca nell'interesse

il medico è esentato sia in sede civile sia in sede penale dal risponderne. Mi sembra francamente un po' troppo!

una parte importante di questo emendamento 7.7 (e mi dispiace che il senatore Malan, forse perché adesso impegnato nel ruolo di senatore Segretario, non sostenga tale in modo particolare, il secondo capoverso, dove si dice: «*Al* *comma 2* *sopprimere* *le parole*: "orientate a cagionare la morte del paziente o comunque"». Vorrei far notare che questo inciso

esattamente il contrario di quanto abbiamo detto prima, e di quanto da voi sostenuto, che il tutto deve essere limitato ad idratazione e alimentazione. Guardate che questo passaggio del comma 2 è assolutamente contraddittorio rispetto a quanto voi stessi avete scritto nella legge.

non ho compreso compiutamente l'intervento del senatore Procacci, ma non vorrei che sembrasse che ho presentato tale emendamento e poi non lo sostengo. L'emendamento lo voterò, ma non posso obbligare altri a votarlo allo stesso modo.

che aveva espresso poco fa la maggioranza, cioè che potessero essere cambiate la terapia o le indicazioni che erano state indicate, se ci fossero stati dei reali cambiamenti

Segnalo soltanto due cose divertenti dell'articolo che stiamo per approvare (noi per la verità cercheremo di respingerlo). È un articolo tutto sulla centralità del medico. Decide lui. Non conta più nessuno: non conta il paziente e in verità, secondo voi, non conta neanche il collegio medico di cui al comma 5, il cui parere non è neanche vincolante per il medico curante, che fa quello che vuole. che il giudice tutelare è invece vincolato ad un parere conforme espresso dallo stesso collegio. Cioè il collegio medico non è vincolante per il medico curante, ma è vincolante per il giudice tutelare. Credo che siamo davvero ad un livello surreale di legislazione, Grazie,

di consultazioni, con l'intervento di una quantità notevolissima di figure specialistiche, per concludere poi che, dopo tutta questa consultazione barocca, il parere resta al medico. Mi chiedo se chi ha costruito questo articolo si sia consultato con chi ha steso il testo della legge sulla semplificazione.

stato ritirato. Onorevoli colleghi, poiché non sono stati approvati emendamenti all'articolo 7 tali da modificarne il contenuto in modo sostanziale rispetto al testo proposto dalla Commissione,

Signor Presidente, ringrazio il presidente D'Alia, che mi concede alcuni minuti per illustrare questa materia un po' particolare, che concerne i dati sensibili. un'illustrazione preventiva, perché tra i lavori di Commissione e quelli d'Aula vi è già stato un accoglimento, da parte della maggioranza, delle indicazioni che avevamo fornite

Sono dati personali che forniscono indicazioni significative in ordine a convinzioni etiche, ideologiche e filosofiche della persona e come tali sono meritevoli della tutela rafforzata, in materia dagli articoli 20 e 26, ovvero 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, del 2003, pena una inammissibile violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza. Ora va sicuramente dato atto che in prima battuta vi è stato un passo in avanti con la riconsiderazione secondo cui questi dati erano considerati non sensibili. Un passo sicuramente positivo è costituito dal fatto che si mira ora a garantire con questa norma, in primo luogo che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sia il solo e unico titolare del trattamento, così da escludere la possibilità di duplicazione di dati da parte di terzi. Fin qui, siamo

debba essere attribuita natura di trattamento, che comporta rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 del codice della *privacy*, al trattamento relativo ai dati contenuti nella DAT, così qualificando tali dati come ipersensibili, in quanto espressivi di quel cosiddetto nucleo duro della identità e della stessa dignità della persona, e per questo meritevoli di una tutela rafforzata in quanto espressivi delle convinzioni profonde della coscienza individuale della persona.

Gli ulteriori emendamenti nella medesima prospettiva propongono in subordine di qualificare i dati contenuti nella DAT quantomeno come sensibili, assicurando così loro tutte le garanzie connesse a tale qualificazione.

che un atto scritto quale è quello che contiene la dichiarazione anticipata, ancorché complesso e con l'assistenza del medico, possa essere oggetto di un intervento di un pubblico ufficiale, ad esempio il notaio. Nessuno può escludere, infatti, che il soggetto interessato e il medico si rechino dal notaio per autenticare le proprie firme, oppure perché si rediga un atto pubblico.

che - trattandosi di atto scritto - ci possa essere questo intervento, attribuisce al Governo la potestà di introdurre nel regolamento

a questo tipo di dichiarazioni e a provvedere anche che questi atti vengano trasmessi nell'archivio tenuto dal Ministero della salute o dalle ASL. Dunque questa

Presidente, vorrei invitare i proponenti a ritirare

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a conclusione di questo faticoso *iter* parlamentare sento di ringraziare tutti i colleghi del Partito Democratico, a cominciare dalla presidente Finocchiaro. Può darsi che sul piano dell'immagine siamo apparsi divisi, anche se il nostro statuto prevede su questioni etiche libertà di coscienza vera. Noi questa libertà di coscienza l'abbiamo realmente esercitata, davvero. Siamo stati autentici e io francamente preferisco l'autenticità

Mi hanno colpito le parole pronunciate ieri dalla senatrice Bianconi, collega stimata e stimabile, la quale diceva: «Abbiamo blindato l'articolo 3, abbiamo chiuso su questo tema», come se fosse ad una riunione del suo Gruppo e non in una seduta del Senato, chiedendo di non modificare neppure una virgola del testo. Le nostre parole sono state altre: sono state ricerca, dialogo, mediazione, sintesi. Parole rifiutate, nonostante i tentativi di mediazione che hanno cercato di portarci oltre la nostra posizione. Questa pagina di incomunicabilità e mancanza di dialogo della vita parlamentare rischia di aprire, signor Presidente, una fase di aspra divisione nel Paese. con conseguenze negative, che non faranno crescere il Paese e la sua unità. Di questo vi assumete la responsabilità

abbiamo discusso per tre giorni, alla fine anche l'intervento del senatore Procacci ha introdotto le dichiarazioni di voto anticipate. Mi sembra che sia un buon auspicio verso il voto finale.

sottosegretario Davico, si è finalmente proceduto ad uno sgombero importante di un campo nomadi nel quartiere San Martino presso Rho, nell'*hinterland* milanese.

preoccupanti, è ora di evidenza generale. Purtroppo queste azioni sono ancora rare ma riteniamo che con il coinvolgimento diretto della cittadinanza che si fa parte attiva e segnala

Signora Presidente, sono nuovo di quest'Aula e lei mi consentirà, quindi, qualche imperfezione nel linguaggio e se dico qualcosa che non è consentito lei mi interromperà subito con il garbo che le è proprio. Desidero sapere se in quest'Aula sia consentito come prassi o da Regolamento che un senatore o una senatrice parli diffusamente all'Assemblea o al Presidente continuando a masticare una gomma americana. Lo chiedo perché vorrei adeguarmi, pensando di passare dal mio tabagismo alla masticatura del tabacco. Se questo ormai, come ho visto, è consentito - e lo è perché nessuno è mai intervenuto

a proposito dei censimenti nei campi rom, che prevedeva una serie di promesse a proposito dell'integrazione, in particolare per i minori e per le scuole. Chiedo di sapere cosa il Governo abbia realizzato a seguito dell'istituzione dei commissari *ad acta* e del censimento. La pregherei di sollecitare una risposta in Aula del ministro Maroni.